"Il link apre una nuova finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

in un convegno dedicato al professor Biagi, ho chiesto di rinnovare anche in questa sede il suo ricordo, in prossimità del quattordicesimo anniversario della morte, per due ragioni. La prima si riconduce all'immanenza della violenza nella nostra dimensione pubblica lungo larga parte della nostra esperienza repubblicana. Oggi temiamo soprattutto il pericolo esterno indotto da un terrorismo che opera su scala globale, ma non possiamo sottovalutare un fenomeno interno, autoctono, che ha già dimostrato di avere caratteristiche carsiche e che si può sempre avvalere di un brodo colturale tutt'altro che assorbito. La seconda si riferisce invece all'attualità dell'intuizione di Marco Biagi, nel momento in cui viviamo la quarta rivoluzione industriale prodotta dalla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Non potremmo altrimenti spiegare il caso, pressoché unico, di un intellettuale nel cui nome si svolgono ancora, dopo molti anni, numerose iniziative che muovono dalla sua visione per analizzare i cambiamenti in atto nel nostro mercato del lavoro ed individuare i possibili percorsi di aggiustamento delle nostre politiche per favorire una crescita accompagnata una crescita accompagnata da un'adeguata intensità occupazionale. Ieri, a Roma, i suoi allievi e una giovanissima generazione di loro allievi hanno sviluppato la sua lezione sostenendo che solo una ancor maggiore delega sussidiaria alla contrattazione collettiva di prossimità e agli accordi individuali certificati potrà consentire l'adattamento delle modalità di svolgimento agile delle prestazioni lavorative ai nuovi moduli organizzativi della produzione di beni o di servizi. ci hanno in particolare ribadito che egli aveva ragione da vendere quando, in un tempo di evoluzione tecnologica molto più lenta, individuava nel diritto all'apprendimento continuo la migliore tutela dei lavoratori rispetto ai pericoli di esclusione sociale. Domani, a Bologna, la Società italiana di medicina del lavoro gli dedicherà le sue riflessioni sui nuovi modi con cui garantire la sicurezza dei lavoratori nel momento in cui l'Internet delle cose o i *robot* rendono obsolete le tradizionali dimensioni aziendali e, in esse, le postazioni fisse, consentendo prestazioni da remoto. Di Marco Biagi sarà ricordato il rifiuto del formalismo giuridico e l'approccio sostanzialista all'obiettivo primario della salute nel lavoro. Contemporaneamente, a Modena, si rinnoverà il periodico seminario internazionale da lui a suo tempo promosso per applicare anche al diritto del lavoro quel metodo comparatista che oggi, ancor più di ieri, consente la convergenza delle regole e delle politiche in un mondo interconnesso. Insomma, signora Presidente, cari colleghi, noi dobbiamo ricordare Marco Biagi per incoraggiare molti giovani a seguire il suo esempio di progettista visionario, di ricercatore curioso che dell'università voleva fare un permanente motore di innovazione, dedicandovisi a tempo pieno con la rinuncia alla libera professione forense. Ambizioso di sapere e di far sapere più che di potere, un vero e proprio maestro di vita. *(Applausi).* Signor Presidente, è sicuramente molto difficile ricordare il momento abbiamo vissuto quattordici anni fa, quando uno studioso di alto livello è stato trucidato per mano di brigatisti, di terroristi che hanno compiuto un gesto violento non solo contro una persona, ma contro un Paese che Biagi voleva provare a cambiare con le sue idee. Marco Biagi collaborava con l'allora ministro Roberto Maroni ed era impegnato in un grande tentativo, quello di modernizzare il mondo del lavoro nel nostro Paese, cercando di introdurre degli elementi di novità che potessero permettere ad un numero più ampio di lavoratori, spesso atipici, di godere di maggiori tutele. Quando si parla di Marco Biagi bisogna parlare delle sue idee, che nonostante tutto hanno continuato a diffondersi, anche nelle Aule parlamentari, ed hanno trovato negli anni un'applicazione concreta. Forse questa è la vera testimonianza della sconfitta di coloro che pensavano di uccidere un uomo e pensavano di uccidere anche le sue idee che, se condivise, avrebbero condotto il nostro Paese verso uno sbocco diverso e sicuramente migliore sotto il profilo occupazionale, favorendo i giovani, ma anche coloro che si trovavano esclusi dal mondo del lavoro in età non più giovane e che sono stati presi in considerazione nelle proposte che ha fatto Marco Biagi assieme ad altri studiosi di valore. Pensare che uccidere un uomo come Marco Biagi potesse arrestare il diffondersi delle sue idee e di un diverso modo di concepire il lavoro, non più legato a retaggi oramai non più funzionali allo sviluppo ed incapaci di attrarre investimenti, è stato un evidente errore, perché le sue idee sono state *humus* per le più evolute teorie giuslavoristiche: anche questa è stata la forza di Marco Biagi. C'è qualcuno che lo ha ricordato un anno dopo la prima commemorazione dalla sua scomparsa: «Nel giorno della commemorazione di Marco Biagi, ad un anno dalla sua tragica morte, è forte la tentazione di rivolgersi ai suoi assassini con le parole che essi meritano, parole di disprezzo senza condizioni, parole prosciugate da ogni lacrima. A dar retta ai sentimenti verrebbe da dire loro: "Chiunque tu sia, dovunque tu ti nasconda, non avrai mai da me né perdono né umana compassione". Ma noi siamo diversi da questi da questi feroci criminali del comunismo armato, per noi il rosso è il simbolo dell'amore, non del sangue innocente che essi vigliaccamente hanno versato. Non dimenticheremo, mai non ci chiedano di provare pietà, ma oggi il nostro pensiero, il nostro ricordo, il nostro affetto sono tutti per la vittima, per le vittime del terrorismo e per le loro famiglie. Per chi ha responsabilità amministrative di governo non c'è migliore modo di ricordare e rendere omaggio al sacrificio di un grande servitore dello Stato che completare il disegno riformatore per cui gli è stata tolta la vita. La sintesi del progetto di Marco Biagi, che egli così sapientemente aveva esposto nel Libro bianco sul mercato del lavoro, è condensata nelle righe finali del suo ultimo editoriale, pubblicato sul «Il Sole 24 Ore» lo stesso giorno in cui veniva brutalmente ammazzato:

Signor Presidente, l'anniversario dell'assassinio di Marco Biagi ci ricorda tragicamente l'ultimo sussulto del terrorismo brigatista. Quel 19 marzo del 2002 rappresentò infatti un terribile salto nel passato, un ritorno a quegli anni di piombo che sembravano ormai appartenere alla storia e non più alla cronaca del nostro Paese. Per il terrorismo rosso i giuslavoristi sono sempre stati i primi nemici, nemici da eliminare in nome di una declinazione estremista e distorta degli interessi della classe operaia. La riforma del mercato del lavoro è stata per troppo tempo un tabù per la sinistra, o meglio, per una parte della sinistra, quella che considerava le riforme il male assoluto. Un mercato del lavoro, quello italiano, che Biagi definì il peggiore dal punto di vista della sua capacità di inclusione, cioè di determinare alti tassi di occupazione, ma che negli ultimi vent'anni, grazie al processo riformatore avviato prima con la legge Treu, poi proprio con la legge Biagi e quindi con il *jobs act*, qualche passo in avanti finalmente lo ha fatto. Ciò è importante ma non sufficiente e il freno maggiore è sempre arrivato dalla parte più conservatrice del sindacato, che fu acerrima avversaria di Biagi e della sua dottrina della flessibilità (la *flexicurity* di cui tanto si parla oggi era l'anima del suo Libro bianco). Eppure, grazie alle politiche ispirate a quella dottrina il nostro mercato del lavoro ha registrato, pur con tutte le sue contraddizioni, una dinamica di crescita ininterrotta per i primi anni del 2000, nonostante le *performance* scadenti dell'economia e un sistema di *welfare* divenuto ormai obsoleto, che usava le risorse dei più deboli a favore dei più forti, ma che nell'immaginario di una parte del Paese si ergeva e si erge come l'ultimo muro di Berlino della sinistra ideologica. La lezione di Biagi, che il ministro Sacconi ha molto ben declinato negli anni di Governo del centrodestra, è molto semplice: l'Italia non andrà da nessuna parte, non riuscirà mai ad affrontare i nuovi bisogni e a riconoscere i nuovi diritti se non sarà in grado di riequilibrare la spesa sociale in favore dei giovani. A quattordici anni dalla morte, Marco Biagi resta dunque il discrimine tra il riformismo di chi sa guardare al futuro e il massimalismo conservatore. Biagi lavorava per un *welfare* che includa, che rimetta in circolazione il lavoro e che non tenda più a escludere, a tenere ai margini i disoccupati, attraverso l'emersione e la trasformazione dei sussidi assistenziali da mera integrazione al reddito, a incentivi per un veloce reimpiego. La grande intuizione di Biagi fu quella di garantire un sostanziale equilibrio tra una maggiore flessibilità di ogni singolo rapporto di lavoro e la maggiore protezione della persona nel mercato del lavoro. Se negli anni Novanta le idee di Marco Biagi sembrarono fin troppo innovative, in realtà rappresentavano un orizzonte necessario che si doveva assolutamente percorrere, a partire dalla creazione di un mercato del lavoro più moderno, più inclusivo, più aperto ai giovani e alle donne, agli esclusi di sempre. Di sicuro, senza la battaglia di Biagi oggi saremmo più indietro nel percorso di modernizzazione del lavoro. Nell'eredità che ci ha lasciato e che i suoi assassini non hanno potuto cancellare, al primo posto c'è il lavoratore come titolare di un accesso pieno e continuo alle conoscenze e alle competenze che, sole, possono garantirgli un posto attivo nel mercato del lavoro e nella società. Tutto questo era al centro del pensiero del grande socialista riformista che oggi ricordiamo con dolore e riconoscenza. Presidente, cosa posso aggiungere a quello che ieri ha detto il presidente Grasso e che hanno detto gli onorevoli senatori questa mattina? Marco Biagi non Marco Biagi non aveva scorta né usava un'auto di servizio. Andava in bicicletta dalla stazione a casa quando ha incontrato i tre brigatisti che gli hanno tolto la vita. Marco Biagi si è imbattuto in una coda del brigatismo rosso che ha insanguinato l'Italia per molti anni e che nel 2002 sembrava già sconfitto. Si è imbattuto in quella coda e nel tentativo velleitario, disperato e criminale di rinverdire quel tipo di terrorismo farneticando del piano del capitale. Devo dire a quest'Assemblea che questo tipo di farneticazione sul piano del capitale che mette a rischio tutte le libertà, i diritti e le democrazie non è nato soltanto dalle menti di piccoli borghesi tentati dal fanatismo; è la conseguenza anche della nostra incapacità di riformare, dei limiti del nostro dibattito politico e culturale già in quegli anni. Le questioni della trasformazione del nostro Paese erano poste nostro Paese erano poste già dalla fine del *boom*, a metà degli anni Sessanta. La classe politica, ma anche la classe dirigente *lato* *sensu* del nostro Paese non le ha affrontate; per questo sono cresciute delle pericolosissime derive come quelle del terrorismo. Marco Biagi rispetto a tutto ciò si proponeva come un ottimo professore di diritto del lavoro e cercava di individuare il cambiamento nella continuità, tentando di non disfare lo statuto dei lavoratori, che porta la firma, tra gli altri, di Brodolini e che è stato un momento alto del dibattito politico e culturale del nostro Paese, ma di adeguarlo alle nuove esigenze.

(forse i meno giovani di voi ricordano la battaglia per abolire la pena di morte in Francia nel 1981), il quale ha scritto un preambolo al nuovo codice del lavoro dove certamente si apre moltissimo alla flessibilità e alle esigenze delle aziende ma

i rapporti di forza e i rapporti fra lavoratori dipendenti e datori di lavoro senza una riforma organica. Lo abbiamo fatto lasciando fare, cioè nello stesso modo con cui abbiamo messo mano alle riforme costituzionali. Davanti alla memoria di Marco Biagi, che ricordo con rispetto, dovremmo allora tutti quanti essere un po' più prudenti e un po' più consapevoli delle nostre responsabilità.

mentre rientrava a casa dopo una delle tante instancabili giornate di studio e lavoro. La settimana precedente un settimanale aveva pubblicato la notizia secondo cui il giuslavorista era nel mirino delle Brigate rosse. Biagi non volle cambiare neanche un piccolo gesto della sua quotidianità (è appena stato ricordato che quella sera tornava a casa dalla stazione in bicicletta), pur sapendo che era minacciata la sua stessa esistenza, andando in giro nella sua Bologna senza scorta. Purtroppo, tornò a colpire quel terrorismo cieco e barbaro che aveva già ucciso insigni studiosi come Ezio Tarantelli, Roberto Ruffilli e Massimo D'Antona, tutti colpevoli di voler modernizzare il mercato del lavoro, realizzando un bilanciamento tra flessibilità e sicurezza e ponendo in campo una serie di contrappesi e garanzie sociali. Il lavoro di Biagi era stato assolutamente trasversale, mettendo le sue enormi qualità di studioso a disposizione dello Stato, in qualità di consigliere dei Governi Prodi, D'Alema, Amato e Berlusconi, consigliere del ministro Maroni, proprio nel momento in cui gli venne tolta la vita. Gli tolsero il bene più prezioso, ma non riuscirono a fermare i suoi studi scientifici e rigorosi, che sono diventati la riforma dell'ordinamento del lavoro in una legge a lui dedicata. Proprio il suo lavoro di studioso del diritto del lavoro di altri Stati più moderni e dinamici del nostro dovrebbe costituire il suo più rilevante insegnamento. I suoi studi, a partire dal Libro bianco, che contiene proposte serie e concrete sul mercato del lavoro in Italia per salvaguardare il potere di acquisto della retribuzione, oltreché il suo valore assoluto, sono un monito quotidiano di fronte a una crisi economica che non accenna a finire; un sistema del lavoro più giusto, che offrisse più opportunità, valorizzasse e premiasse il merito e portasse con sé prospettive e programmi: Marco Biagi era abituato a immaginare il futuro. È necessario ricordare la sua importante opera, che deve diventare un patrimonio condiviso, così come è importante avere come esempio duraturo e quotidiano la sua figura di uomo. rivolgere un ultimo pensiero alla signora Biagi e al figlio Lorenzo, che hanno dovuto subire la perdita di un grande uomo, sottratto dalla più spaventosa e ignobile vigliaccheria di chi preferì sparare spesso alle spalle degli indifesi.

è legata da un filo profondo che, ancora adesso, a quattordici anni dal tragico assassinio, ci invita ad approfondire e ad attingere al suo pensiero, oltre che per ricordarne la figura umana, anche per affrontare il presente e progettare il futuro. Il coraggio di compiere scelte, di progettare soluzioni nuove, basate su un'attenta analisi delle dinamiche e dell'incongruità del presente era la base culturale di uno studioso che amava definirsi "giurista a progetto" e che, tra i propri motti preferiti, aveva il significativo «progettare per poter riformare». Il saper affrontare le tematiche del mercato del lavoro in un'ottica non provinciale, ma attenta alle dinamiche internazionali, era all'origine del metodo comparativo portato avanti da Marco Biagi, ripreso dal suo maestro, il professor Mancini, dettato dalla profonda convinzione che - sono parole di Biagi - «solo chi conosce le esperienze di altri sistemi giuridici può valutare quanto avviene nel proprio ordinamento interno. La comparazione non è semplice esercizio culturale. Si tratta invece di comprendere approfonditamente le ragioni che hanno portato a certe soluzioni piuttosto che ad altre». La comparazione - proseguiva Biagi - «è l'unica prova di laboratorio di cui dispone il giurista». Un metodo che permetteva a Biagi di uscire dai fortini consolidati dei giuristi formalisti e gli rendeva abituale il confrontarsi a tutto campo, anche con gli attori politici, sociali ed economici, in un'ottica interdisciplinare e dinamica, non conoscendo ambiti autoreferenziali o rigidità ideologiche. Su questa base egli ha dato un grande contributo alla legislazione del lavoro, a partire dal suo Libro bianco e dal suo recepimento nelle successive leggi, fino al tragico momento dell'assassinio.

per la prima volta la moglie Marina prese la parola in pubblico, intervenendo di fronte ad un'ampia platea di ragazzi e ragazze delle scuole bolognesi, senza mai andare sopra le righe e con delicato dolore. Disse allora Marina: «Dopo che persone infami lo hanno ucciso, il suo nome è stato associato alla precarietà: questa è una bugia terribile. Marco al contrario voleva proteggere chi si sarebbe trovato in questa situazione di difficoltà».

non un corpo di norme a sé stante, ma un intervento organico, progettato fin dai tempi della collaborazione con il primo Governo Prodi, per estendere i livelli di tutela a tutte le forme di lavoro. Lo Statuto dei lavori - scriveva Biagi - «dovrebbe finalmente dare all'Italia nuove tecniche per regolare tutti i tipi di lavori, anche quelli più atipici, rivedendo vecchie norme non più in sintonia con la moderna organizzazione del lavoro e prevedendone delle nuove capaci di governare i mestieri emergenti...». Come non vedere qui l'anticipo di quel giusto statuto del lavoro autonomo che proprio in queste settimane sta uscendo? Come scriveva Biagi nel 2002, il mercato e l'organizzazione del lavoro si stanno evolvendo con una velocità non paragonabile a quella del passato e l'orizzonte nazionale non è più sufficiente a delineare, da solo, le regole del diritto del mercato in questa crisi globale, i suoi insegnamenti continuano, per contemperare i valori dell'efficienza con l'equità, della competitività con la coesione sociale; obiettivi che danno un'anima e una precisa direzione ad una parola troppo spesso usata solo come slogan: la *flexicurity*. Impegnarsi a fondo per combattere le vere "precarietà" del nostro mercato del lavoro, seguendo ed aggiornando questi insegnamenti, è la migliore risposta sia all'atto barbaro che ci ha privato di Marco sia alle tante polemiche strumentali e superficiali che hanno ingiustamente offuscato la sua figura dopo.

ho ascoltato con attenzione quanti sono intervenuti nella discussione generale di ieri sul tema dell'istituzione di questa giornata per la commemorazione delle vittime innocenti della mafia. Come mi aspettavo, non ci sono state voci contrastanti.

come credibilmente incontra il sentire della stragrande maggioranza dei cittadini italiani, ovvero di tutti quelli che fanno riferimento alla legalità come metodo di vita sociale. Il fatto che tutti siano concordi sull'istituzione di questa giornata, mi ha però sollevato un dubbio e mi ha fatto accendere

cittadini italiani si sentono a rischio nel momento in cui denunciano, perché ancora oggi perché ancora oggi sono sotto la pressione della criminalità organizzata, che ha trovato, in un'alleanza con lati oscuri della grande impresa del nostro Paese, degli elementi di sinergia. saluto con giusto entusiasmo questo disegno di legge,che ho immaginato possa costituire una sutura tra la società civile, che lotta contro la mafia, e lo Stato, che si mette correttamente alla sua testa. al tempo stesso rivolgermi a tutti noi, che abbiamo responsabilità di rappresentanza politica, e al Governo, che ha la responsabilità della gestione delle Forze dell'ordine e delle azioni sociali a contrasto di tutte le storture e di tutte le mancanze e le carenze della società,

Signora Presidente, colleghi senatori, si conclude oggi un percorso avviato su iniziativa di vari senatori appartenenti a diversi Gruppi parlamentari. Saluto positivamente questa conclusione e la convergenza che si è determinata su questo testo. È importante che venga approvato un disegno di legge che ha l'obiettivo di esaltare la memoria delle vittime innocenti di mafia,

È ormai sempre più evidente che non bastano più le sole azioni di polizia o le sentenze emanate dalla magistratura. Ogni giorno le cronache ci segnalano i risultati dell'intensa e proficua attività di contrasto esercitata dalle forze di polizia e dalla magistratura, che ringrazio, perché quei risultati sono il frutto di una grande capacità investigativa, di una grande dedizione al lavoro e anche della capacità di grande coordinamento tra le diverse forze di polizia e tra le istituzioni dello Stato. Allo stesso modo, ogni giorno vengono segnalate le attività che si concludono attraverso l'emanazione di misure di prevenzione di natura patrimoniale, che costituiscono sicuramente

occorre l'impegno e il protagonismo dei cittadini, perché venga diffusa e praticata la cultura della legalità, perché ciascuno si senta titolare di diritti da rivendicare con ogni forza, piuttosto che

una capacità di esercizio del controllo del territorio e delle attività, anche di natura istituzionale, attraverso l'uso della corruzione: sempre più evidenti risultano le relazioni tra attività criminali esercitate da organizzazioni mafiose e camorriste e l'uso della corruzione. È quindi che venga richiamato l'impegno non solo delle istituzioni, ma anche dei cittadini, per liberare la società dal dominio criminale. Questo vale sicuramente nelle tante realtà del Mezzogiorno dominate dalla forza criminale, ma anche per le realtà più ricche del Paese, sempre più insidiate dalla penetrazione criminale, mafiosa e 'ndranghetista. È necessario essere consapevoli di quanto sia opportuno e determinante aggiornare le politiche e le azioni di contrasto. Occorre mettere in campo nuovi strumenti, capaci di rendere impenetrabili i meccanismi che regolano la vita economica, sociale e le attività delle istituzioni repubblicane. Noi assumiamo ogni giorno questo orizzonte e pensiamo che la nuova cultura antimafia debba essere accompagnata dall'impegno a rendere sempre più efficiente e trasparente il meccanismo di funzionamento delle istituzioni pubbliche, solo la trasparenza, solo la tracciabilità delle decisioni e delle attività di natura pubblica e la partecipazione diretta dei soggetti interessati, anche attraverso la contrapposizione di interessi divergenti, può garantire l'esercizio democratico e liberale nelle attività economiche e nelle attività sociali. Serve quindi una robusta cultura democratica e la consapevolezza che attraverso il rispetto delle regole e l'esercizio della legalità i problemi che abbiamo di fronte

Grazie

i due momenti centrali di una giornata che ci impegniamo tutti a far diventare un grande momento della vita del Paese, in grado di scuotere le coscienze e di rinnovare l'azione contro le mafie che, com'è stato detto, ha bisogno sia del momento della memoria, sia dell'altro importante momento dell'impegno. Nel momento dell'impegno bisogna costruire una nuova dimensione progettuale della stessa antimafia tale progettualità rientrano le università, le associazioni nazionali antimafia impegnate ed un cammino nuovo che l'antimafia deve percorrere con umiltà, correggendo anche gravi errori

in modo assolutamente leale, nel rispetto delle leggi e adempiendo al proprio dovere è un ostacolo importante all'infiltrazione della criminalità mafiosa,

Il titolo del disegno di legge recita: «Istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie».

la definizione di «vittime della mafia», secondo la quale: «Per vittime della mafia si intendono le persone fisiche decedute o che hanno riportato lesioni a causa di eventi di matrice criminosa di stampo mafioso. Sono altresì vittime della mafia anche le persone giuridiche che hanno subito atti da parte della criminalità organizzata di stampo mafioso. In entrambi i casi il riconoscimento dello *status* di vittima della mafia non può prescindere dall'esser estraneo a tale ambiente criminale».

Grazie E non a caso, questa modifica è subentrata perché la Giornata del ricordo delle vittime della mafia ha subito una trasformazione nel senso di quella che è la definizione stigmatizzata dall'associazione Libera. Come Libera ha introdotto il termine innocenti, siamo andati ad aggiungerlo anche noi. Le iniziative noi. Le iniziative parlamentari qui dentro sono poche o nulle, perché noi ci occupiamo di conversione dei decreti-legge. Tuttavia, le poche leggi che abbiamo affrontato non sono di iniziativa parlamentare, ma provengono dalle varie associazioni:

al taglio dei vitalizi dei parlamentari, voluto sempre da Libera, che effettua queste pressioni. Ma il nostro Senato potrà o no tornare ad avere una propria sovranità,

giornate commemorative, che ieri sono diventate 254 e quando approveremo la giornata del dono, anche quella frutto di una pressione esterna, diventeranno 255:

Senatore Calderoli, lei dice che questo emendamento sarà bocciato, però non sarà respinto con i voti del mio Gruppo perché noi lo votiamo e per una ragione semplice, anzitutto di ordine linguistico, perché il concetto di vittima include in sé la condizione di innocenza. È molto difficile immaginare

di seguire le indicazioni che vengono da soggetti estranei alla politica, sostenute attraverso loro rappresentanti che fanno di quella attività

Io non ci sto, noi non ci stiamo e diciamo ciò che riteniamo giusto dire, a prescindere dai suggerimenti. Questo Senato non deve accogliere suggerimenti da parte di alcuno, se non da parte del popolo italiano.

di rottura di questa unione che si dovrebbe realizzare nel giorno in memoria delle vittime della mafia. Immaginate solo per un istante se, per ipotesi, si aprisse una discussione, un dibattito, tra vari comitati o associazioni che siano, perché su tre morti ammazzati dalla mafia, forse il terzo non è una vittima innocente:

l'impegno di tutti contro la mafia, educando alla legalità. Questo ovviamente contraddice l'ipotesi che la vittima fosse un mafioso. Se fosse un mafioso non sarebbe vittima della mafia.

non c'è un giudice, non c'è un processo, non c'è un'autorità che potrà stabilire quali sono le vittime innocenti e quali no. È evidente, invece, che potrà essere da tutti condiviso che il mafioso, ossia colui che è condannato per rapporti con la mafia

senza avere alcuna colpa, un atteggiamento ostile. Addirittura, la vittima era quella sacrificale, il capretto portato al sacrificio. È inutile aggiungere la parola «innocente», quindi appoggio questa ripulitura del testo, che mi sembra solo di buonsenso. Signora Presidente, raramente sono d'accordo con le posizioni espresse dal senatore Calderoli, però devo dire che questa questione La qualificazione di innocente è all'interno della qualificazione di vittima, in quanto la vittima non può che essere innocente; altrimenti è partecipe di un'azione che ha sicuramente connotati di negatività, senza arrivare all'omicidio o alla violenza fisica. Da questo punto di vista, quindi, invito il relatore

più che il ricordo o la memoria noi dovremmo mettere in campo l'impegno e l'impegno ha bisogno di quotidianità, non di ricordo o di attività in un'unica giornata dell'anno. Tra l'altro, non credo che il nostro Paese abbia bisogno di normative che richiamino la memoria; ha bisogno di provvedimenti legislativi - senza eccedere, per la verità che programmino il futuro, che indichino obiettivi concreti, che affrontino i problemi che l'Italia e gli italiani hanno. Cerchiamo di lasciare il ricordo agli archivi delle associazioni - meritorie, per carità - e di soggetti che vogliono garantirsi una visibilità politica attraverso una iniziativa legislativa di questo genere spazio a un impegno più concreto e più difficile, che è quello della individuazione dei percorsi per dare a questo nostro Paese una prospettiva che ha difficoltà ad individuare. Signora Presidente, è intervenuto il senatore Caliendo per il mio Gruppo quindi, evidentemente, giustifico il mio intervento con il voto in dissenso. Pregherei l'Assemblea di fare attenzione. State riducendo questa Giornata della memoria a un fatto squisitamente giuridico. State legalizzando un valore.

quelle finalità sono tutte tese alla costruzione di una cultura dell'antimafia, sono tutte tese al ricordo dei fatti eclatanti della storia e della cronaca di questo Paese, che prescinde purtroppo - ahimè - dal dettaglio delle singole vittime e porta la discussione e il confronto sul complesso delle vittime, su quanto di atroce un'organizzazione criminale è riuscita a fare in questo Paese. Ma davvero voi pensate che in una manifestazione all'interno di una scuola si parlerà del figlio di Di Matteo, che è vittima della mafia, pur essendo il padre mafioso? Si parlerà di altro. Davvero voi credete che in quelle manifestazioni vi sarà un ricordo vero e reale di quello che precedette l'omicidio di Giovanni Falcone e la sua vicenda, tutta interna al mondo giudiziario e che portò, ahimè, della magistratura a non indicarlo in Commissione come procuratore nazionale antimafia? Se volete istituire un giorno della memoria - e sono d'accordo con voi - non potete che prescindere dai dettagli e scrivere «innocente» è un dettaglio, perché, come è scritto nelle preleggi, nella interpretazione della legge i lavori preparatori sono importanti, il testo della legge è importante e nei lavori preparatori a nessuno è venuto in mente di scrivere che tra le vittime della mafia vi è anche il mafioso ucciso dai suoi consociati mafiosi. E a nessuno è venuto in mente di scrivere nel testo che quelle manifestazioni dovranno avere ad oggetto questo e non qualcosa di più alto. Nella ricerca dell'unanimità all'ennesimo disegno di legge di istituzione di un giorno della memoria, credo che dei dettagli dobbiamo fare a meno, perché se quei dettagli portano acqua al mulino dell'associazione che magari li ha suggeriti, non portano davvero acqua all'unanime votazione di un provvedimento simbolo e di un provvedimento giusto. Non posso votare a Non posso votare a favore essendo intervenuto in dissenso dal mio Gruppo e quindi mi asterrò. Ma di certo dico che, se deve restare il termine «innocente» all'interno del testo,

per certi versi non posso che apprezzare, perché se veramente inauguriamo una stagione in cui prestiamo attenzione alla qualità della tecnica legislativa e alle parole che possono essere più o meno utili all'interno delle nostre norme, forse d'ora in avanti riusciremo davvero a produrre norme più efficaci e meno equivoche. vorrei esprimere le ragioni per le quali, dopo aver meditato a lungo, ad esempio nel disegno di legge a mia prima firma, abbiamo condiviso l'idea di mantenere la parola «innocenti». Vorrei dire - lo dico con grande

è affermare che ci sono tante vittime innocenti: ci sono bambini, di uno o due mesi, che hanno perso la loro vita semplicemente perché si sono trovati nel posto sbagliato in un certo momento, Grazie

i familiari delle vere vittime della mafia ci hanno chiesto di fare nostra, e hanno lavorato affinché tutti noi dessimo un contributo per la cultura della legalità, e non dall'antimafia, anche se ovviamente la cultura dell'antimafia è importante,

come ha detto qualcuno - che distinguano chi è innocente da chi non lo è (ci sono già degli organi a ciò preposti), mentre c'è bisogno di riaffermare che ci sono tante persone che lavorano affinché coloro che vogliono verità e giustizia sociale siano riconosciuti anche dal Parlamento. Grazie

di benefici previdenziali a favore delle vittime della mafia, introducendo una fattispecie. Oggi, per legge, rischiamo di creare una dicotomia rispetto a quella che per me è una posizione singola, unitaria e unica: le vittime della mafia non possono che essere vittime innocenti. Se uno è vittima della mafia e lavora per la mafia è un criminale,

vuole essere un ricongiungimento tra la lotta contro la mafia effettuata da elementi importanti della società civile e lo Stato che, come ho detto, si mette alla guida, com'è giusto che sia, di questa battaglia. La dicitura «vittime innocenti» è quello che la società civile ha prodotto e sedimentato in tutti questi anni. È sicuramente una qualificazione più etica che giuridica, come giustamente ha fatto rilevare il presidente Calderoli. Ritengo comunque che abbia un suo significato. Tutto ciò premesso, non voglio sprecare la possibilità che tutta l'Assemblea si esprima in modo univoco su questo provvedimento, perché è estremamente importante che ciò

Grazie

Presidente, ovviamente gli ordini del giorno sono stati presentati prima della votazione in Aula e io ho riportato quanto previsto nel testo base in discussione,

era una giornata di primavera - precisamente dieci giorni dopo l'equinozio del non troppo lontano 1984 quando a Nardò, un Comune come tanti del mio Salento, una giovane donna amministratrice, l'assessore alla cultura e alla pubblica istruzione, Renata Fonte, veniva freddata in modo atroce, con gesto vigliacco, da tre sicari sull'uscio di casa. La giustizia, in questo caso, ha fatto il suo corso. I colpevoli sono stati arrestati e gli assassini sono stati condannati.

Renata è oggi, non solo in Puglia, sinonimo di speranza per la politica locale: una politica e una responsabilità che meritano qui una digressione in ragione dei dati sempre più preoccupanti che riferiscono di una crescita esponenziale delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali e su cui attendiamo la relazione finale da parte della Commissione di inchiesta istituita proprio in Senato. Renata è anche esempio per i giovani, che possono trovare nella sua pur breve vita un valido e autorevole modello cui ispirarsi, un riferimento valoriale e comportamentale. È dunque nel mese di marzo (il mese che, per antonomasia, associamo alle donne e che le celebra nel mese della primavera) che si dà vita ad un'iniziativa che intende seminare e diffondere quei sani anticorpi che nascono, si sviluppano e crescono con la memoria storica condivisa in difesa non solo delle istituzioni democratiche, ma anche del senso primo e nobile della libertà della persona. Abbiamo impresso nella nostra mente il principio per il quale le idee camminano sulle gambe degli uomini e delle donne che si rendono e si prestano ad essere i loro pratici esempi. A tal proposito, quest'oggi il mio pensiero è rivolto anche ai ragazzi incappati in quella che appare come un'insopportabile beffa del diritto e che dovrebbe raccogliere in quest'Assemblea l'attenzione di noi tutti.

che, riuniti da anni in una cooperativa, gestivano, dopo averlo rimesso in sesto, un *resort* confiscato al *boss* Sorangelo. Ebbene, dopo dodici anni di processo e a vent'anni dai fatti contestati, la Corte d'appello di Bari ha annullato tale confisca, rimettendo nel possesso del Sorangelo questa struttura, nonostante le evidenti irregolarità. È una storia amara, questa, con un bruttissimo epilogo,

che auspico diventi legge a breve, occorre narrare i «successi dello Stato nelle politiche di contrasto e di repressione di tutte le mafie». Per tali motivi, dichiaro il voto favorevole e convinto al provvedimento

L'argomento oggi in discussione richiama un tema che ha animato la ricerca nelle più svariate discipline, dalla sociologia alla biologia, dall'antropologia alla filosofia. Solo per citare quest'ultima, duemila anni di speculazione intorno alla memoria hanno animato filosofi come Platone, Sant'Agostino, Leibniz e Spinoza, fino ad interessare storici come Le Goff, che rappresentano soprattutto il nostro tempo. Cito Le Goff non a caso, perché ne riparlerò fra un attimo. Un tema fascinoso ed importante, insomma, che forse avrebbe meritato ben altro tempo e ben altra considerazione (ma tant'è) e che conseguentemente ci impone almeno due domande: cos'è la memoria? Cos'ha di così importante la memoria? La memoria altro non è che la capacità di ricevere, conservare e recuperare informazioni: archiviazione e rievocazione. Ma la memoria può essere di diversi tipi, può essere individuale, collettiva, biologica, storica, culturale e nella nostra epoca anche robotizzata. E che cos'ha di importante la memoria? Ha - anche secondo il vecchio adagio latino *historia lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae* - il merito di ricordare che è inevitabile che, se si dimentica il passato, si ripetano gli stessi errori. Occorre invece tenere viva la memoria storica da una generazione all'altra, perché il passato non si ripeta allo stesso modo. Bene, ciò premesso, quello che il disegno di legge in discussione oggi chiede è l'istituzione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Perché abbiamo bisogno di questo? Solo per rievocare? Certamente È perché abbiamo bisogno di trasferire dei valori, abbiamo cioè ritenuto che il lavoro, l'opera, la vita, l'impegno e la testimonianza delle vittime che andiamo a ricordare rappresentino dei valori che vanno tutelati e salvaguardati. Ritorno allora al citato Jacques Le Goff, che scriveva: «Storia e memoria si nutrono l'una dell'altra, ma non si confondono tra loro». Questo era ed è un monito, perché la storia è ed è stata di fatto troppo spesso manipolata, per dare legittimazione ideologica ai poteri politici e per celebrare le loro glorie nascondendo le loro nefandezze. È il caso nostro questo? Assolutamente no. Ma continuava Le Goff: «A fianco della storia manipolata dai vari poteri bisogna continuare a costruire un sapere storico fondato sulla ricerca della verità». E a noi questa verità storica cosa ci dice? Questa tremenda verità storica del sacrificio di tante vittime innocenti di mafia cosa ci dice? Ci dice che il loro sacrificio è stato vano; il Paese è marcio in ogni ordine e grado. L'altro ieri, sul «Corriere della Sera», in modo molto mirabile lo ha testimoniato il costituzionalista Ainis, quando ricordava del politico milanese arrestato mentre andava alla giornata della trasparenza, quando ci ha ricordato del quando ci ha ricordato del paladino della lotta al *racket* condannato per estorsione, o quando ci ha ricordato del magistrato icona delle ecomafie che il CSM ha sospeso per i suoi rapporti con i *clan*. Per le corruzioni dilaganti all'ANAS, per quelle nella Guardia di finanza e nelle commissioni tributarie e - aggiungo io - per lo spettacolo sconfortante delle primarie del PD, per l'insensata scelta di candidare Bertolaso, imputato di corruzione, a sindaco di Roma. E poi ancora - di questo ne sono testimone - ci sono anche i tre anni in quest'Aula, dove la violazione di norme e regole è stata la norma. Alla luce di tutto questo, a me viene da chiedermi e da chiedere: abbiamo - e mi ci metto dentro anch'io, insieme a tutti quelli che non hanno potuto usufruire del beneficio di inventario - la legittimazione morale per chiedere quello che stiamo chiedendo? stiamo chiedendo? Uso le parole di don Ciotti, che amabilmente avete riportato nella prefazione al disegno di legge: «Non possiamo limitarci a ricordare, per quanto il nostro dovere sia di non dimenticare. Dobbiamo trasformare la memoria in impegno, denuncia, testimonianza e cambiamento». Abbiamo queste credenziali? Io credo proprio di no. So che poi arriverà il nel concetto di «*omnia munda mundis»*, ma come Conservatori e riformisti non possiamo stare a questo gioco e non permetteremo che la vita, la storia, il lavoro e il sacrificio di valenti uomini dello Stato o di sconosciuti cittadini italiani diventi la foglia di fico sotto la quale, a poco prezzo, potrete lavare la vostra coscienza. Noi ci asterremo da questa votazione. Signora Presidente, abbiamo già assistito a qualche intervento, riguardante anche l'esame degli emendamenti, su cui abbiamo molto apprezzato la posizione del Governo e dell'Assemblea.

l'istituzione di una giornata nazionale della memoria e dell'impegno per ricordare le vittime delle mafie è sicuramente un dato positivo. Ogni giorno, nel nostro Paese, c'è una storia da ricordare: una storia intrisa di dolore, che racconta di vite spezzate e spazzate via dalla mano vile di chi utilizza la violenza per ottenere vantaggi personali, in modo prepotente e illegale. storie di uomini e donne che hanno scelto di stare dalla parte della legalità, pagando un prezzo altissimo. Voglio fare una chiosa anche per i familiari, che hanno vissuto tali situazioni. Ogni giorno è un riaffiorare di dettagli e di ricordi che uccidono ancora: nomi, fotografie, articoli sui giornali, processi nelle aule dei tribunali. Storie di una quotidianità, di famiglie, di affetti annullati per sempre. È un dovere morale, per chi resta, mantenere viva la memoria di chi non c'è più, ma lo è ancora di più per le vittime di mafia. Diventa una sorta di "urgenza'", per i familiari delle vittime, mantenere viva almeno la memoria di chi è stato ucciso in nome della dignità, dell'onestà e per affermare la legalità. Questa giornata servirà a far vergognare esecutori materiali e mandanti, servirà a trasmettere un po' di forza e di coraggio ai tanti magistrati che ogni giorno subiscono tutte le difficoltà della lotta contro la criminalità organizzata

pulita questa nostra società dal cancro delle mafie. Sono state circa 1.120 le vittime innocenti di mafia che hanno

e della tracotanza mafiosa. Sono le storie di coloro che si sono battuti e sono stati ammazzati, di quelli che hanno avuto il padre sbagliato o che hanno parlato troppo e dei tanti altri ammazzati o colpevolmente dimenticati. Ci sono

che la mafia cadesse sotto i rigori del codice penale, come associazione criminale. La mafia ha massacrato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, da vivi hanno inflitto alla mafia colpi risolutivi, capaci di dare alla lotta antimafia sviluppi che in precedenza non era neanche possibile ipotizzare. Da morti hanno animato un movimento antimafia di massa, che ha cambiato la realtà di questo Paese. Nella lotta alla mafia, va da sé che il modo in cui la si combatte deve essere sempre il più ampio possibile. Ci sono doveri pubblici e doveri privati, ci sono doveri individuali e doveri collettivi, doveri sociali e doveri istituzionali. Giovanni Falcone sosteneva che la mafia è un fatto umano che ha avuto un inizio e avrà anche una fine e starà a noi cercare di capire quando sarà, il prima possibile. La mafia è fatta di organizzazioni mutevoli, capaci di evolversi, di cambiare pelle con il cambiare delle epoche, di celarsi camaleonticamente nelle pieghe e nelle zone grigie della società. La lotta alla mafia è diventata un impegno quotidiano, costante, esclusivo e totalizzante; impegno che non ammette nessun ripensamento né tentennamento, una scelta di vita da portare avanti con spirito fermo e determinato, consapevoli di rischiare la vita, l'emarginazione e l'isolamento. è la condizione che ha accompagnato i vari Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Giuseppe Di Lello e Leonardo Guarnotta. Tommaso Buscetta, un attimo prima di iniziare a svelare ai giudici i segreti dell'organizzazione criminale più potente del mondo, aveva detto: la avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà una celebrità, ma cercheranno di distruggerla, fisicamente e professionalmente. Non dimentichi che il conto che lei ha aperto con Cosa nostra non si chiuderà mai. Signor giudice, è sempre del parere di interrogarmi? la risposta fu affermativa, un sì dettato dalla certezza e dalla consapevolezza che la mafia è come un parassita che consuma la società e la vita degli individui, che si attacca come una sanguisuga a qualsiasi attività che produce denaro. una differenza rispetto a un comune parassita: mentre certi parassiti infestano le loro vittime e le consumano fino a farle morire, la mafia è un parassita intelligente, intelligente, che lascia alla sua vittima quel tanto di nutrimento che le serve per sopravvivere e quindi per continuare a produrre per lui, per succhiare indisturbata il sangue della società sana di questo Paese, soprattutto il fiume di denaro che scorre nei grandi appalti. Di questo la mafia è capace. chiare manifestazioni della forza intimidatrice tipica del potere mafioso. Abbiamo visto in TV alcune scene raccapriccianti. Dopo la vita, il bene comune più prezioso che le organizzazioni mafiose mettono in pericolo e danneggiano è certamente la democrazia.

negli anni, inoltre, i nostri esperti antimafia hanno sempre sostenuto che la migliore lezione di legalità e quindi di antimafia è far funzionare questa Repubblica: tanto meglio funziona la Repubblica, quanto meno c'è bisogno di mafia. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa disse che lo Stato avrebbe battuto la mafia quando avrebbe assicurato come diritti ciò che i mafiosi elargivano come favori. Dall'altra sponda, quella mafiosa, ci sono le parole del boss Pietro Aglieri, che disse sostanzialmente ad un magistrato: vede, dottore, quando voi andate nelle scuole e parlate ai vostri ragazzi, quelli vi ascoltano, ma quando escono e cercano un lavoro chi trovano? Trovano noi La storia ci dice che la memoria è molto importante e l'impegno nel ricordo lo è altrettanto (parlavo proprio d'impegno prima, signor Presidente), ma vanno entrambi tenuti vivi. Come sapremmo dell'Olocausto se a raccontarlo fosse stato il boia e non il deportato n. 174517? Ciò vale per la vittima innocente della mafia, del terrorismo e di ogni grande

non condividiamo le conclusioni cui è giunto il senatore Di Maggio, che ha dichiarato il voto di astensione del suo Gruppo,

Grazie

si consuma nel nostro quotidiano, con le nostre azioni di ogni giorno e ciascuno di noi sa come conduce il proprio quotidiano e quindi ciascuno di noi sa se ha o no tale legittimazione. Spero che il mio

Vedete, la storia recente ci ha insegnato che l'organizzazione mafiosa e le organizzazioni criminali

quando nascevano dei moti popolari, delle organizzazioni spontanee di contrasto alla mafia,

è stata illustrata da noti studiosi e giornalisti che hanno analizzato il fenomeno della criminalità organizzata e in particolare della mafia. Quindi che cosa pensarono di fare? Pensarono di fare propri questi moti e dunque, nel giro di poco tempo, nacquero decine, centinaia di associazioni antimafia. La dimostrazione che questa analisi è corretta sta nel fatto che molti soggetti, anche nel mondo della politica, hanno utilizzato e strumentalizzato tali associazioni per fare carriera politica. Io vedo sindaci che fanno indossare la striscia tricolore ad una donna vittima della criminalità organizzata, magari durante la processione di una festa patronale, e poi leggo che quella stessa amministrazione comunale, diretta da quel sindaco, è condizionata dalla criminalità organizzata. l'eroina dell'antimafia, così definita dalla stampa e dall'immaginario collettivo del territorio siciliano,

Io avrei preferito un disegno di legge che avesse introdotto nelle scuole, come esisteva una volta, la materia educazione civica. In quel tempo, forse, vi era la necessità di educare i bambini a delle condotte che fossero civiche. Oggi non c'è più questa necessità, ma avrei preferito l'introduzione di una materia che educasse alla legalità. Sarei stato più soddisfatto, perché avrei fatto qualcosa di più concreto. Oggi noi approviamo questa norma, che istituisce la Giornata della memoria.

sconfiggere la mafia e la criminalità organizzata? Io credo di no. È un provvedimento simbolico, ma, nella sostanza, quando in Campania, la mia terra,

Napoli), questo soggetto è immediatamente bersaglio della criminalità organizzata, nel senso che viene acquisito alla propria organizzazione. Quando lo Stato è assente e una organizzazione di diversa e di qualsivoglia natura si sostituisce ad esso, quella organizzazione attecchisce. Noi abbiamo in quest'Aula diversi studiosi della criminalità organizzata. Mi riferisco alla senatrice Capacchione che, con sobrietà, ha sempre svolto il suo lavoro di attenzione al fenomeno della criminalità, e della camorra in particolare.

creare quei presupposti e quei germogli di crescita della criminalità organizzata. È in quella direzione che noi dobbiamo andare. Non dobbiamo soltanto limitarci a dire al ragazzo di ricordarsi delle vittime della criminalità e della mafia. Noi dobbiamo dare ai giovani del nostro Paese anche una prospettiva di futuro e di vita, in un alveo della legalità. Se non facciamo questo, ci trasformiamo in quel genitore

quel figlio non gli darà ubbidienza, perché non gli riconoscerà l'autorevolezza di dargli ordini, disposizioni e regole.

importante e positivo. Non da oggi sosteniamo la tesi che la memoria sia un elemento decisivo nell'educazione civile di una popolazione, soprattutto in un Paese come il nostro, così segnato e scosso in tutti questi anni dal fenomeno della criminalità. Ci pare di poter dire che il provvedimento che ci accingiamo a varare stamattina si pone fortunatamente in continuità con quelle parti più attive, più significative e anche più vive di esperienze sociali e civili in tutti questi anni hanno avuto il merito straordinario di tenere sempre la porta aperta - se così e di non far dimenticare mai quello che dovrebbe essere sempre il punto di riferimento anche di quest'Assemblea parlamentare. Non dobbiamo commettere l'errore di pensare Grazie

anzi riconoscere che, anche dal punto di vista della politica, probabilmente nel corso di questi anni quella soglia di attenzione, che pure in una fase particolarmente emotiva della storia di questo Paese - per esempio, a metà degli anni Novanta, dopo la morte di Falcone e Borsellino in particolare - era ovviamente molto elevata, purtroppo con il tempo si è abbassata. Credo che questo sia un monito per tutti quanti noi. C'è stata una fase in Italia, appunto, nella quale, anche sulla scorta di una grande emotività popolare, la politica e le istituzioni, lo Stato, i partiti, hanno saputo insieme fare quadrato e mettere in campo processi di autoriforma e processi legati alla necessità storica di battere un colpo e di segnare un elemento di frattura e di discontinuità. Credo che quella soglia di attenzione, che pure in anni non lontani è stata molto alta e significativa, il tempo purtroppo si sia abbassata, come se davvero avessimo fatto l'errore di pensare che la battaglia era vinta, e che, per l'appunto, la vittoria di quella battaglia ci consentiva di abbassare la soglia di attenzione. Forse abbiamo riflettuto e abbiamo indagato poco, o almeno non sufficientemente, sul fatto che invece le mafie si trasformavano con grande velocità e grande capacità, dal loro punto di vista anche con grande efficacia, sotto i nostri occhi; sul fatto connotazioni sempre diverse rispetto al passato, sempre più pervasive. Ci siamo detti spesso, anche all'interno di quest'Aula parlamentare - e abbiamo fatto lo stesso anche nelle Commissioni preposte, in particolare nella Commissione antimafia quanto fosse necessario mettere in campo un ragionamento che sapesse riconoscere le nuove mafie: mafie fatte spesso non più di immagini classiche, non più di

mettere in campo una strategia di contrasto altrettanto efficace di quella che lo Stato seppe mettere in campo quindici anni fa.

il contrasto alle mafie e alle criminalità organizzate debba essere vissuto esattamente con la stessa intensità con cui tanti anni fa le giovani generazioni di questo Paese

non dobbiamo mai dimenticare (e ce lo dicono proprio quelli che più di tutti si sono battuti in questi anni per tenere vivo il ricordo delle vittime innocenti della criminalità)

Signora Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che oggi trattiamo e che stiamo per approvare mi coinvolge direttamente e personalmente da siciliano. Ricordo ancora quando, quarant'anni orsono, superato l'esame di maturità, arrivai nella città di Palermo per iscrivermi all'università. Ricordo cos'era Palermo Personalmente, poteva capitare di camminare nelle strade del centro - non nelle desolate periferie - finanche in piazza Politeama o davanti al teatro Massimo e assistere a scene incredibili. Quando non si assisteva a scene incredibili, spesso si udiva nel centro della città il tragico rumore delle armi da fuoco. Io stesso ricordo - e talvolta mi sovviene con terrore durante la notte - il rumore terrificante dei*kalashnikov* che vennero usati per la prima volta contro le vetrine di una nota gioielleria del centro, per effettuare una tragica prova balistica (era la prima volta che arrivavano quelle armi in Sicilia), per poi procedere a un numero enorme di omicidi. Sappiamo tutti cosa rappresenti, in termini di male assoluto, la mafia in Sicilia, la 'ndrangheta in Calabria, la camorra in Campania, la sacra corona unita in Puglia e tutte le mafie nel resto del Paese e anche al di fuori dei confini nazionali. Sappiamo cosa hanno prodotto in termini di devastazione, di disegualità, di devastazione (uso ancora questo termine) delle coscienze, della socialità in termini di diseconomia. Sappiamo tutti quanto sia lungo l'elenco delle vittime, iniziando dal 1893 (omicidio Notarbartolo) dal 1909 (omicidio Petrosino). È una serie infinita di vittime e di omicidi. Ricordare tutti i nomi sarebbe quasi impossibile e supererebbe non soltanto il tempo a mia disposizione, ma quello di tutti i Gruppi parlamentari. Ma alcuni nomi vanno ricordati: il procuratore Scaglione, Peppino Impastato, Piersanti Mattarella, Pio La Torre, Carlo Alberto Dalla Chiesa e la moglie Emanuela Setti Carraro, Rocco Chinnici, Fava, Rosario Livatino, Giovanni Falcone con la moglie Francesco Morvillo, Paolo Borsellino, gli agenti delle loro scorte, l'avvocato Famà e altri ancora. Come poi non ricordare la tragica e lunghissima serie di sindacalisti ammazzati

Casarrubea, Placido Rizzotto, Spagnolo, Bongiorno e il mio concittadino Accursio Miraglia, trucidato a Sciacca il 4 gennaio 1947. Fino ad oggi abbiamo lasciato all'iniziativa delle comunità locali, degli enti locali e delle associazioni il ricordo ogni anno delle vittime della mafia, un ricordo che serve a tenere vivo nel nostro Paese la memoria, affinché si sviluppi una coscienza che in ogni cittadino, in ogni ragazzo e in ogni giovane faccia sorgere forte la volontà di dire no e di opporsi con determinazione a tutte le mafie. Sappiamo come ogni anno il 21 marzo, primo giorno di primavera, giorno che leghiamo alla memoria di San Benedetto e quindi alla rinascita dell'Europa e del mondo allora civile rispetto alla barbarie delle invasioni e dell'oscurità seguita alla caduta dell'impero romano, Libera celebri la giornata della memoria e dell'impegno, il ricordo delle vittime innocenti della mafia. Dal 1996, ogni anno, in una città diversa, viene letto un elenco di circa novecento nomi di vittime innocenti. In quell'elenco ci sono nomi che ci danno subito un'emozione fortissima; ci sono delle vittime il cui nome ci dice poco, vittime sconosciute ai più. Ma proprio per questo, è ancora più forte il dovere di ricordarle tutte unendole in un unico tragico filo rosso di sangue, di violenza, di terrore. Quest'anno la giornata si svolgerà a Messina e, in contemporanea, in tanti luoghi del nostro Paese. E la giornata del ricordo delle vittime, che come dicevo si svolgerà all'unisono su tutto il territorio nazionale, come sempre come sempre consentirà di rendere vivo il ricordo di quei nomi, di quei sacrifici, di quei martiri. Di fronte a un fenomeno così importante, che coinvolge, scuole, istituzioni, associazioni, i familiari delle vittime e i singoli cittadini, credo che vada accolto con grande soddisfazione il lavoro svolto dai colleghi in Commissione affari costituzionali e il lavoro che oggi stiamo qui svolgendo con un voto che mi auguro più ampio possibile, perché questo è un provvedimento che merita, nell'interesse del Paese - e uso questa espressione forse un po' aulica e desueta - una grande condivisione. Con questa legge in tutto il territorio nazionale, presso scuole, università, tribunali, enti territoriali e in tutte le istituzioni, si potranno svolgere iniziative, anche in collaborazione con forze dell'ordine, con la magistratura, con associazioni imprenditoriali, antiracket e antimafia, dirette proprio a far nascere e coltivare nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni la memoria delle vittime della mafia, ciò che rappresenta la loro storia. È giusto che non si dimentichi, e soltanto con l'istituzionalizzazione di tale giornata si sancirà un'altra tappa dello Stato nella lotta contro la mafia. ha già raggiunto grandi risultati: l'arresto dei latitanti, la disarticolazione dell'organizzazione su vaste parti del territorio, la confisca dei beni, l'evidenziare zone grigie di contiguità, l'istituzionalizzazione nel nostro codice del 41- *bis*, il codice antimafia, l'istituzione del fondo unico giustizia. Sono tutte cose già fatte. Ma è ancora più importante non soltanto fare queste cose, segnali segnali che la politica ha già dato, ma soprattutto sottolineare come l'antimafia sia diventata e possa ancora rappresentare un valore unificante e caratterizzante della nostra identità nazionale. Si stabilisce quindi che in tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in occasione della giornata, si promuoveranno, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia e delle vittime della criminalità organizzata. Emerge chiaramente, signora Presidente, come tali iniziative rappresenteranno quindi non soltanto una mera occasione celebrativa, ma l'opportunità per riflettere, approfondire e discutere di un problema purtroppo ancora attuale e, soprattutto, si ha la fondata speranza di potere contribuire a promuovere tra gli studenti e tra i giovani il sentimento della legalità e di appartenenza ad una patria che accomuna tutti cittadini attraverso valori condivisi. Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono ormai trascorsi più di venti anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio

e soprattutto far conoscere questa storia e queste radici ai giovani. Chi non ha memoria del proprio passato è destinato ad un incerto futuro e proprio noi siamo convinti con determinazione che questa giornata della memoria contribuirà a far nascere e a far crescere una nuova generazione di italiani. È per questo che convintamente il Gruppo al quale appartengo, il Gruppo di Area Popolare, Nuovo Centro Destra e UDC, voterà convintamente questo disegno di legge. Signora Presidente, vorrei iniziare questo intervento dalle seguenti parole: «La mafia - affermava Antonino Caponnetto, procuratore della Repubblica teme più la scuola che la giustizia», dal momento che «l'istruzione toglie l'erba sotto i piedi della cultura mafiosa». Questo è stato l'*input* che mi ha spinto a depositare la proposta di legge che è stata oggetto di esame congiunto con la proposta della senatrice Dirindin che discutiamo oggi. Sono trascorsi, ormai, più di venti anni dalle stragi di Capaci e di via D'Amelio e, per poter combattere la cultura mafiosa e le sue manifestazioni più o meno estreme, è necessario innanzitutto avere contezza della storia e delle sue radici, e soprattutto farle conoscere ai giovani. Se la memoria è fra i pochi valori capaci di nobilitare e salvare dalla quotidianità della vita, troppo spesso tuttavia dimentichiamo di rievocare e onorare quelle figure esemplari che hanno segnato in modo indelebile la storia del nostro Paese, figure come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino che, accomunate dal tragico destino di vittime della mafia cui si erano fieramente contrapposti, hanno rappresentato entrambi un'icona indiscussa di legalità, onestà e coraggio. Troppo spesso le nuove generazioni rimangono all'oscuro anche del più recente passato e, dunque, senza sapere neppure chi siano stati Falcone e Borsellino e cosa abbiano rappresentato. «Gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini», sosteneva Falcone. Ma, affinché ciò possa verificarsi, non si deve dimenticare il sacrificio di questi umili servitori dello Stato. Le loro idee dovrebbero risiedere nella coscienza civile e nel lavoro di tutti coloro che, opponendosi alla prevaricazione e all'eclissi delle coscienze, scelgono ogni giorno il valore dell'onestà. Riteniamo fermamente che Falcone e Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992, rappresentino l'emblema della legalità e della lotta civile alle organizzazioni criminali. Essi raffigurano - anche visivamente - la *ratio* che intendevamo perseguire con il disegno di legge presentato, ovvero conservare e costruire una memoria storica delle vittime innocenti delle mafie, nonché i successi della magistratura che opera in difesa delle istituzioni democratiche. La legalità va di pari passo con la conoscenza e la responsabilità: accrescere una cultura della giustizia e della legalità permette, dunque, di responsabilizzare studentesse e studenti, stimolandone le coscienze. Permettetemi di dire che riconoscere una giornata nazionale della memoria per le vittime della mafia come atto in sé - a mio avviso - non ha alcun significato se non viene effettivamente concepita e programmata come momento di riflessione e di ricordo con iniziative concrete. Ora, nell'evidenziare l'approvazione di un nostro emendamento che richiede agli istituti scolatici di ogni ordine e grado la promozione di iniziative volte alla sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia, dobbiamo anche constatare che la nostra specifica proposta di invitare gli stessi istituti scolastici a esporre un'immagine di Falcone e Borsellino, il cui valore è anche quello di contribuire a non dimenticare, purtroppo non è stata accolta, ma è stato accolta dal Governo e dal relatore sottoforma di ordine del giorno. È chiaro che l'affissione di un'immagine è un atto simbolico, nel rispetto dell'autonomia scolastica, che tuttavia riteniamo molto importante e carico di significati perché rappresentativo di un'icona indiscussa di legalità, onestà e coraggio che, proprio negli ambienti scolastici, dovrebbe essere evidenziata. Questa era davvero la *ratio* che doveva avere il disegno di legge in esame. L'iniziativa, unitamente agli eventi di sensibilizzazione e di riflessione comune, non costituiscono solo un'occasione celebrativa ma un'opportunità per riflettere, approfondire, discutere, per promuovere tra gli studenti quel sentimento di legalità e di appartenenza a una stessa Patria che dovrebbe accomunare tutti i cittadini. Per quanto fin qui detto comunico a quest'Aula il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle.

si pensa a una sola organizzazione criminale ed è sbagliato. Una delle prime ragioni per cui voterò, con tutto il Gruppo di Forza Italia, a favore del provvedimento è che correttamente si parla di mafie al plurale, ossia di quelle organizzazioni criminali che sono presenti in varie parti del nostro Paese. Basta solo ricordare che la Regione Lombardia, in cui vivo, ha indicato la necessità di una giornata di memoria come quella che stiamo votando. Queste organizzazioni criminali si atteggiano e si pongono con le stesse caratteristiche che contraddistinguevano per alcuni anni, almeno agli occhi di chi la percepiva, la mafia siciliana. Ma era un errore limitarsi solo a questo. Il relatore - correttamente, devo dire - esordisce nella sua relazione con le parole: «L'educazione alla legalità costituisce un valore». È questa la logica che Rocco Chinnici aveva presente ogni volta che ragionava di dover andare in tutte le scuole. Io andavo tutti i mesi a Palermo per incontrarlo, essendo stato responsabile della sua nomina. Egli andava nelle scuole perché riteneva che l'intervento giudiziario non avrebbe mai risolto il problema delle mafie. Occorreva un'educazione alla legalità, che non vuol dire soltanto rispetto delle leggi. Leggendo

con le varie autorità per favorire amici e parenti e, quindi,

Borsellino, di essere stata loro vicina, o aver contribuito a determinati sviluppi dell'azione della magistratura contro la mafia,

Giovanni Falcone era un civilista e non aveva mai fatto un giorno di penale, essendo occupato nella sezione fallimentare prima a Trapani e, poi, a Palermo. Tuttavia, proprio applicando le regole del civile e seguendo il percorso del denaro, riuscì a fare il grande processo a Cosa nostra,

Delle persone oneste. Infatti, basterebbe leggere i distinguo, le precisazioni, le valutazioni e le votazioni al Consiglio superiore della magistratura

a un livello tale da indurre un rifiuto spontaneo, radicato e convinto dei metodi delle organizzazioni mafiose.

che diventa difficile un'azione della magistratura. Quindi, è necessario lo sradicamento dall'interno delle nuove generazioni, educate a dei valori che siano tali da non essere più condivisi quando vengono avvicinati da organizzazioni diverse, che gli prospettano quanto meno un possibile guadagno facile.

l'emendamento che abbiamo votato, ne ho fatto una questione proprio perché si ispirava a questa logica. La logica è: chi è mafioso non è vittima, chi partecipa alla cultura mafiosa non è vittima. È vittima chi si comporta nella legalità, la quale - come ho detto prima - non è solo il rispetto della legge penale. Penso a quelli che sono a mezzo viatico tra l'uno e l'altro, quelli che, per propri interessi personali, inducono le persone a credere che vi sia la possibilità di ottenere qualcosa attraverso metodi all'apparenza legali,

ma anche al metodo elettorale. Se la legge elettorale non garantisce una rappresentanza effettiva e proporzionale delle minoranze, vuol dire che non è una democrazia effettiva. su questo che dovremmo tentare di ragionare insieme, sperando di poterlo fare nelle scuole, perché solo così lasceremo ai nostri figli un'Italia diversa, un'Italia in cui sarà condannato dalla magistratura chi sbaglia. Ma non avrà alcuna responsabilità lo Stato per non aver garantito una situazione tale da consentire a chi vuole vivere nella legalità di vivere con la libertà.

a partire dalla Presidente, che ringrazio per l'attenzione e l'impegno profuso nei confronti del provvedimento in esame. Pur trattandosi di un piccolo provvedimento, di una piccola goccia in un settore che ha bisogno

In primo luogo è il momento della memoria e dell'impegno, perché la responsabilità e la cultura della legalità partono anche dal ricordo, dal rispetto e dall'impegno che ne possono derivare, con riferimento alle vittime innocenti delle tante mafie che in questo Paese intervengono quotidianamente nel funzionamento dei nostri sistemi.

la presenza delle mafie sul territorio nazionale. Noi non facciamo che riconoscere un'esperienza importante, che si è costruita negli ultimi venti anni e che è cresciuta in maniera significativa. Vorrei dare qualche elemento di conoscenza rispetto a questa esperienza, che molti di noi conoscono e forse qualcuno soltanto in parte. - viene celebrata il 21 marzo, perché è il giorno in cui si esce dal lungo buio e dal freddo dell'inverno e inizia una stagione nuova, che risveglia la natura - vuole essere il culmine di un percorso molto lungo, dalle associazioni dei familiari, dai gruppi, dalle scuole e da molte delle organizzazioni che operano almeno dal 1996, per ricordare le vittime innocenti delle mafie.

quali sono gli interventi che possono essere messi in campo, con senso di responsabilità e impegno, affinché le istituzioni democratiche non possano essere ulteriormente indebolite.

la quantità di giovani, i quali, quando si parla di legalità, partecipano e si impegnano in maniera gioiosa, ma con grande senso di responsabilità.

I giovani, rispetto alla legalità, mettono in campo iniziative, energie e disponibilità, per discutere e preparare il 21 marzo,

per capire che cosa vuol dire cultura della legalità; per capire perché le mafie si infiltrano nella pubblica amministrazione e nell'economia; perché riescono a condizionare il comportamento delle persone e, soprattutto, perché non dobbiamo rassegnarci.

sa cosa voglia dire vedere decine di migliaia di persone in silenzio che ascoltano per due ore l'elenco delle vittime della mafia: lo fanno con rispetto e dignità, pronti subito dopo a realizzare iniziative sempre per ricostruire la cultura della legalità.

Nel 2009 una giovane ragazza della scuola di Scampia, quando si preparava il 21 marzo a Napoli,

per impegno o purtroppo per il caso. Il primo problema è dimostrare che c'è un'Italia che non si rassegna, che vuole fare rete, che vuole costruire delle sinergie culturali, politiche, organizzative per promuovere la cultura della legalità

Credo che questo provvedimento dovrebbe aiutarci a riflettere affinché non si continui con quello che è stato denunciato da molti in questa sede come un atteggiamento retorico o semplicemente di denuncia di quanto effettivamente stiamo osservando nei lunghi anni in cui abbiamo ricostruito la storia delle vittime delle mafie. Non c'è bisogno di denunciare: a questo pensano già le istituzioni preposte. Come Parlamento abbiamo il dovere dovere - come stiamo facendo - di raccogliere un'iniziativa che è partita e cammina con le gambe dei familiari delle vittime delle mafie.

se le mafie esistono, se le mafie condizionano i mercati, se le mafie si infiltrano nella pubblica amministrazione e fanno affari a danno dell'interesse generale - dobbiamo dircelo con molta franchezza - è perché noi non glielo sappiamo impedire. Ognuno di noi non sa fare rete, costruire sinergie e impegnarsi effettivamente per impedirlo. perché noi glielo permettiamo, perché la comunità non ha sufficiente capacità di contrastarle, di combatterle e di contrapporre l'integrità, la buona gestione dentro la pubblica amministrazione e l'interesse generale rispetto all'interesse particolare o addirittura all'interesse di una piccola parte che vuole imporre ad ogni costo il suo modo di ragionare. È per questo che abbiamo bisogno più attenzione a questi temi. Non dobbiamo pensare che basti approvare questo provvedimento. Dobbiamo ricordarci ogni giorno che abbiamo approvato un provvedimento

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 98, 248 e 1832.

soggetto, Primo Greganti, frequentava questo Palazzo, chiedo immediatamente una verifica degli ingressi.

Presidente, colleghi senatori, il disegno di legge «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale» rappresenta una tappa importante della stagione di riforme in atto nel nostro Paese, regolando e incentivando uno tra i fenomeni di maggior rilievo cresciuto nel nostro Paese: appunto, il terzo settore. Gli enti di terzo settore concorrono, come già ben chiarito all'articolo 1, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e occupazione. Qui vi è già il primo elemento da sottolineare. Quest'espressione, terzo settore, nei passati trent'anni e fino ad oggi è stata una categoria sociologica o economica, prevalentemente ad uso di studiosi e operatori. Con l'approvazione del disegno di legge diventerà una categoria giuridica. Sono di terzo settore le organizzazioni che rispondono a determinate e precise caratteristiche, e solo a chi dimostra di possederle la legge riconoscerà incentivi e facilitazioni, affinché i vantaggi ricadano a favore dell'intera società. In questi trent'anni di rapido sviluppo il terzo settore è stato disciplinato attraverso normative settoriali, che hanno senz'altro avuto il merito di inquadrare e sostenere fenomeni di grande valore - pensiamo al al volontariato, alla cooperazione sociale, all'associazionismo di promozione sociale - ma lo hanno fatto in modo disorganico, ciascuna norma interessandosi solo di un particolare tipo di organizzazione, talvolta originando inquadramenti giuridici e trattamenti fiscali tra loro non sovrapponibili

delle dita della mano e della mano: finora abbiamo riconosciuto le singole dita. Ora riconosciamo la mano, fatta da più dita ma che fanno parte della mano, capace di muovere in modo coordinato le dita. A fronte di ciò, il Governo circa due anni fa ha avviato l'*iter* legislativo con l'obiettivo di costituire un quadro giuridico sia civilistico sia fiscale che consenta di dispiegare al meglio le potenzialità del terzo settore rendendo la normativa più organica e coerente, di semplificare le procedure, di rendere di rendere più efficaci le azioni di vigilanza e controllo tese a prevenire abusi e scorrettezze. Il lavoro svolto presso la Camera ha contribuito in in modo decisivo all'esito oggi presentato, ponendo stabili fondamenta alla normativa, mentre il lavoro fatto in Commissione affari costituzionali al Senato è intervenuto in modo significativo su molti aspetti che saranno di seguito qui richiamati brevemente e che credo rendano ancora più chiara, coerente ed equilibrata la norma che portiamo oggi alla discussione in Aula. Veniamo ora agli aspetti principali del disegno di legge. Nell'articolo 1 sono definite le caratteristiche del terzo settore: l'assenza dello scopo di lucro, il perseguimento di finalità civiche e solidaristiche di utilità sociale, la realizzazione di attività di interesse generale. nell'azione volontaria e gratuita, nel codice della mutualità e nel codice della produzione e dello scambio di beni e servizi. A partire da tale definizione, il Governo è impegnato con la delega ad approvare i successivi decreti sui più importanti temi: la revisione degli enti di cui al libro I del codice civile; il riordino e la revisione complessiva delle disposizioni relative agli enti di terzo settore, compresi gli aspetti fiscali e tributari; la revisione della disciplina in materia d'impresa sociale; la revisione della disciplina in materia di servizio civile. La delega riguarda anche il sistema delle verifiche, dei controlli e del monitoraggio degli enti di terzo settore, e prevede la dotazione di significative risorse. Con riferimento al lavoro svolto presso il Senato, il Governo si è a questo proposito impegnato, in aggiunta a quanto già previsto nel testo uscito Un'altra modifica riguarda la previsione di disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni. Quanto ai settori di attività, il testo ha modificato la versione proposta dalla Camera e fa un passo avanti nella razionalizzazione della questione, delegando il Governo a giungere ad un unico testo unificato delle attività di interesse generale, appunto un elenco unico che, oltre a rappresentare un elemento di semplificazione, va nella direzione di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, la cui non sovrapponibilità rappresenta un aspetto di complicazione dell'attuale ordinamento. Ciò non esclude che, poi, il Governo possa individuare, sulla base delle vocazioni delle diverse famiglie di terzo settore, ambiti di attività specifici per alcune di esse. La delega, poi, prevede la necessità di approfondire gli aspetti fiscali, oggi caratterizzati da troppe norme, spesso specifiche per ciascuna forma giuridica, rispetto alla quale sarà necessario cercare soluzioni di grande semplificazione. Sempre tra gli interventi proposti in seconda lettura, ve ne sono alcuni a tutela dei lavoratori: ad esempio, l'obbligo di informazione e la necessità di garantire negli appalti pubblici condizioni economiche non peggiorative rispetto a quelle previste nei contratti siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il testo in discussione oggi introduce, poi, una modifica della delega in termini di affidamenti al terzo settore, richiamando le direttive comunitarie. Si introduce un'importante previsione tesa a riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello. Ancora, nell'articolo che riguarda le attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, sono previste tre importanti modifiche. In primo luogo, la previsione di uno specifico riconoscimento e di una valorizzazione per le organizzazioni di volontariato; in secondo luogo, la costituzione la costituzione del Consiglio nazionale del terzo settore, con il superamento degli osservatori nazionali ed una ridefinizione dei compiti attribuiti ai centri di servizio per il volontariato,

l'articolo che riguarda l'impresa sociale, perché ha portato significative innovazioni rispetto al testo già molto preciso che la Camera ci ha consegnato. La discussione all'interno della Commissione ha portato a prevedere che l'impresa sociale rientri pienamente nel complesso degli enti di terzo settore, adottando tutte le caratteristiche proprie di questo

Rispetto alla disciplina degli utili, il lavoro del Senato specifica che la soglia di remunerazione coincide con quella prevista per le cooperative a mutualità prevalente ed esclude che questa eventuale, pur limitata, distribuzione di utili possa essere applicata ai soggetti del libro I del codice civile. Anche questa è stata una decisione molto controversa, ma che ha trovato - credo - un punto di chiarezza definitivo. Anche con riferimento al servizio civile universale sono state introdotte tre importanti modifiche rispetto al testo uscito dalla Camera. La prima riguarda la riaffermazione, che trova le radici nella storia dell'obiezione di coscienza, del servizio civile nazionale come connesso alla difesa non armata. In secondo luogo, il Senato risolve positivamente il problema, più volte oggetto di sentenze in tal senso, dell'apertura del servizio civile agli stranieri regolarmente soggiornanti. Terzo, viene prevista la centralità dello Stato nella programmazione del servizio civile. Con riferimento al tema fiscale, la modifica più significativa riguarda la previsione di una revisione complessiva della nozione di ente non commerciale. Tutto ciò va nel senso di affidare al Governo, come ho già ricordato, il mandato per superare quella che non ho difficoltà a definire una vera e propria giungla di norme fiscali, che appare sempre meno sostenibile. importanti sono anche le dotazioni previste, con nuovi fondi, rotativi e non. E voglio citare in particolare il nuovo fondo, inserito nel testo del Senato, destinato esclusivamente ai soggetti del libro I del codice civile. Si propone inoltre, attraverso un emendamento che il Governo sta per presentare, di istituire la Fondazione Italia sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di adeguate risorse finanziarie (soprattutto private, voglio sottolinearlo) e con il contributo e l'apporto di elevate competenze gestionali, di sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi. Questi ed altri meno importanti sono i cambiamenti che il lavoro della Commissione porta oggi all'attenzione di quest'Aula. Nel complesso sono convinto che il risultato che portiamo alla discussione dei senatori sia di assoluto rilievo, un grande passo avanti nel quadro normativo, che non si limita alla fotografia dell'esistente ma ha l'ambizione di essere traino di una "fase due" del terzo settore.

Per concludere, al terzo settore, a quel popolo di milioni di persone che ogni giorno in Italia si battono, spesso in modo silenzioso, per il bene comune va la mia e - ne sono sicuro - la riconoscenza di tutta l'Assemblea e la nostra ammirazione. La loro volontà, le loro fatiche, la loro intelligenza, la loro compassione prescindono dalle leggi, che siano buone o meno buone. Ma altresì sono convinto che a quel popolo, e a tutto il popolo italiano, potrà arrivare il nostro aiuto, ciò che possiamo fare qui in questi giorni: una legge quadro più chiara, più semplice, facilmente applicabile, con una visione nitida, nitida, capace di promuovere e favorire cittadinanza attiva, coesione sociale, benessere dei cittadini e delle comunità. Io sono convinto che la proposta che discutiamo possa e potrà farlo. Grazie Comunico che è stata presentata una questione pregiudiziale. Ha chiesto di intervenire la senatrice Stefani per illustrare la questione pregiudiziale

Ricordiamo ancora l'articolo 76 della Costituzione per cui la funzione legislativa non può essere delegata se con determinazione di principi e criteri direttivi e per oggetti assolutamente definiti. Noi riteniamo che l'ampiezza della delega, come prevista nella legge, metterà il Governo nell'impossibilità

non essendoci l'indicazione del criterio direttivo, non si comprende dove si potrà andare a verificarne il rispetto dei suoi limiti.

Cosa significa «significante»? È un termine assolutamente generico, perché il significante potrebbe essere di una minima rilevanza. Ma qual è l'indicazione della rilevanza?

ciò che è ancora più pericoloso, perché qui non vi è il limite di una delega; a questo punto, se l'opzione viene lasciata al Governo, non si può che ritenerla un'amplissima delega in bianco.

in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è, per definizione, la legislazione su delega». il Governo delegato non ha dei vincoli, non stiamo più parlando di una legge delega, ma stiamo dando un potere smisurato all'attività governativa. A nostro avviso poi - questo è da aggiungere - i termini stessi previsti per l'esercizio della delega sono privi di univocità. Nascono problematiche, a nostro avviso, proprio per il mancato rispetto degli stessi articoli 114 e 117 della Costituzione, perché quando viene chiesta l'intesa il Governo e la Conferenza unificata, ai fini dell'adozione di decreti legislativi, non viene nemmeno indicato su quali materie sarà necessario acquisire tale intesa. Se non sono indicate le materie, come si farà a individuare i limiti nel decreto? Quali

che il tema del servizio civile sia completamente sganciato dal contesto del disegno di legge delega, con una totale disomogeneità anche di contesto. contesto. All'articolo 2, in cui si enunciano i criteri e i principi direttivi generali, non si fa nemmeno riferimento al tema della revisione del servizio civile.

Questo lo diciamo anche nel merito: vi sono dei problemi, perché non si riesce a comprendere la natura giuridica della stessa iscrizione del registro. Ha un effetto costitutivo? È una pubblicità e quindi ha solo un effetto conoscitivo?

in dubbio se presentarla, anche alla luce di quello che è accaduto in Commissione: abbiamo, da una parte, una legge delega molto filosofica nei suoi principi e, allo stesso tempo, indeterminata che, però, contiene se è venuto meno durante il dibattito in Commissione - l'unico articolo dispositivo, l'articolo 9-*bis*, su cui è stato presentato un emendamento in Commissione da parte del Governo. L'emendamento, alla luce delle riflessioni e degli interventi svolti, spesso anche da esponenti della maggioranza, avrebbe richiesto una riformulazione e poi è stato ritirato per avere una fase evolutiva in sede d'Assemblea.

lo Stato deve metterci un milione di euro tanto per partire. Vorrei allora che per ciascuna *start-up* che esiste in questo Paese e che abbia natura privatistica, come dovrà avere questo soggetto, lo Stato mettesse un milione di euro.

Però, oggi non stiamo discutendo nel merito e invito il Governo a riflettere bene prima di presentare e usare trucchetti vari per poi far passare in Assemblea quello che in Commissione

scrittura da parte del Governo. L'articolo 118, comma 4, della nostra Costituzione recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»; l'argomento dovrebbe essere caro agli amici del centro e della sinistra (più o meno del centro). Una cosa però è chiara: facendo un soggetto del genere, abbiamo una centralizzazione o, meglio, un esproprio un esproprio dell'iniziativa pubblica o privata del terzo settore e di quel mondo che si è sviluppato spontaneamente sul territorio, che in un colpo solo verrebbe centralizzato e, purtroppo, privatizzato, sicuramente non a titolo gratuito.